Successivamente, il ministro dello sviluppo economico, onorevole Bersani, interverrà sulle questioni mafia-imprenditoria siciliana, fabbisogno energetico e andamento dei prezzi dei prodotti alimentari. Ricordo che un senatore per ciascun Gruppo può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda. Dopo la risposta congiunta da parte del Ministro, ciascun interrogante può a sua volta replicare per non più di tre minuti. La RAI ha assicurato la ripresa diretta televisiva per un'ora e mezza. La Presidenza confida nella cortesia dei senatori che interverranno per primi affinché sia consentito al maggior numero di colleghi di intervenire nel corso della diretta.

Certamente non bisogna avere paura dei *media*, che sono attraversati da un cambiamento tecnologico incessante, quotidiano e tuttavia occorre minimizzare i rischi e accrescere le opportunità. Il Governo, anche con per l'uso consapevole dei *media* nel rapporto tra bambini e Internet, ma forse occorre un salto di qualità. Chiedo cosa intende fare il Governo per sensibilizzare maggiormente i genitori, le famiglie e i ragazzi sull'uso consapevole di Internete se anche nella scuola non siano previste

Signor Presidente, signor Ministro, nella precedente legislatura, fu costituito, d'intesa tra il ministro Gasparri e la Commissione bicamerale per l'infanzia, il Comitato "Internet e minori", assolutamente volontario e gratuito,

Il Comitato ha pubblicato un Libro bianco di grande interesse: che fine ha fatto questo libro, che poteva essere veramente uno strumento di guida? Infine, intende il Ministro cercare un'intesa

Signor Presidente, per un giovane Internet è uno splendido strumento di conoscenza, socializzazione, divertimento, studio, creatività, ma le esperienze possibili della Rete, le nuove identità e i ruoli delle esperienze virtuali espongono i bambini, più di ogni altro, ai pericoli di cui la Rete è intessuta. Mi riferisco specificatamente alla diffusione della pedopornografia, di materiale pedopornografico in cui i bambini e le bambine sono vittime due volte: prima, come soggetti sviliti e usati per immagini inimmaginabili; poi come inconsapevoli fruitori dell'orrore, incontrato per caso navigando o ricercato

cerca di tenere insieme il contrasto alla diffusione telematica della pedopornografia e l'esigenza di garantire la libertà di comunicazione e manifestazione del pensiero. La mia domanda è quale sia stato l'esito dei primi sei mesi di monitoraggio effettuato dall'applicazione della normativa che lei ha voluto darci.

di violenza e sopraffazione. Rammentando che proprio oggi il Governo ha aperto il dibattito per la costruzione di una Carta dei diritti della Rete, vorrei chiedere quali sono le strategie del Governo per contrastare il diffondersi su Internet di messaggi di violenza, sopraffazione e pedopornografia e se è possibile l'utilizzo della Rete in modo alternativo, soprattutto in ambito scolastico.

le cronache recenti sono giustamente piene di terribili casi di abusi sessuali, violenze e maltrattamenti in danno di minori. Negli ultimi tempi, queste vicende risultano nascere sempre più spesso nella sfera delle persone che ruotano attorno al minore, sia che si tratti di educatori sia di componenti del nucleo familiare. A questa già drammatica situazione oggi si aggiunge un altro pericolo, vale a dire Internet, che facilmente può essere usato come esca per attrarre bambini innocenti in storie di abusi e loschi traffici. Chiedo, quindi, di sapere quali sono i risultati prodotti dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e se il Governo non ritenga opportuno, nell'ambito delle attività dello stesso Osservatorio o con la costituzione di un'apposita Commissione interministeriale, procedere allo studio di uno specifico Protocollo d'intesa, che coinvolga, procure, prefetture, questure, scuole e servizi sociali per l'adozione di interventi coordinati nell'attività di prevenzione e contrasto al fenomeno, come già sperimentato a Milano.

Signor Presidente, credo che, come tutti i senatori interroganti hanno sottolineato, ci troviamo di fronte a una delle contraddizioni tipiche del nostro tempo. Da una parte, siamo in presenza di una straordinaria macchina di libertà, una straordinaria occasione di informazione, come la Rete;

Al tempo stesso, questa straordinaria macchina di libertà, che porta - come si dice in gergo - un po' il mondo nelle nostre case, perché dà la possibilità alle famiglie e ai ragazzi di avere una quantità di informazioni incredibile rispetto alle generazioni precedenti, alle generazioni precedenti, contiene, come spesso accade, anche dei rischi fortissimi. Quindi, è ovvio che la comunità internazionale e i Governi, perché la questione ha una dimensione globale, devono lavorare per preservare la libertà (se ne sta parlando, come ricordavate, proprio qui a Roma, in un incontro promosso dal Governo, avente come occasione per rafforzare i diritti di libertà) e, al tempo stesso, tutelare le minoranze, le fasce più deboli, in modo particolare i bambini e i minori. Credo che questa minaccia per le fasce

libertà, altrimenti rischiamo d'ingenerare in una parte dell'opinione pubblica e delle nostre famiglie una reazione contraria, che comincia a vedere nella Rete più gli aspetti negativi e i pericoli che non le occasioni positive.

interattività, cioè la circostanza che i bambini, i ragazzi producono contenuti nella rete, attraverso l'*uploading*, è addirittura esploso solo negli ultimi due o tre anni. Quindi, oggi non c'è solo da fare attenzione ai contenuti che arrivano nella Rete in generale, ma anche ai contenuti autoprodotti spesso dai minori e che circolano nella Rete. Che cosa si può fare? Il primo tema su cui credo che i Governi debbano impegnarsi e su cui il nostro Governo, così come i precedenti, è impegnato, è il tema della pedopornografia (ne parlavano le senatrici Valpiana e Pellegatta e il senatore Barbato) come sapete - è una delle minacce più insidiose. Infatti, i siti sono difficilmente individuabili, la loro allocazione è transnazionale,

quindi una minaccia piuttosto pericolosa di cui l'ONU e l'Unione Europea si stanno occupando. Il nostro ordinamento giuridico, come sapete, tutela i minori contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale con la legge la legge n. 269 del 1998. Questa legge è stata integrata nel 2006 con disposizioni più specifiche che riguardano lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo di Internet. Questa norma ha previsto l'istituzione, da parte del Ministero dell'interno, di un Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, sotto la responsabilità della polizia postale e delle comunicazioni. In questo ambito, l'8 gennaio scorso, il mio Ministero ha adottato, d'intesa con il Ministero per le un decreto nel quale, dopo un lavoro fatto con gli Internet *service provider*, si sono individuati gli strumenti tecnici di filtraggio che consentono di intervenire molto rapidamente per oscurare i siti che vengono individuati. Il decreto obbliga i fornitori di connettività a dotarsi di sistemi in grado di oscurare entro sei ore entro sei ore dalla comunicazione ricevuta i siti che diffondono questo materiale. Si è attivato in questo modo un circuito positivo in cui i *provider*, in collaborazione con la polizia postale e delle comunicazioni, effettuano le operazioni per oscurare i siti. Ritengo che questo lavoro abbia prodotto finora risultati operativi molto importanti, che non cancellano naturalmente la minaccia, la quale ha le caratteristiche che dicevo prima: è transnazionale e rispunta sempre in altre forme appena si interviene per reprimerla. Voglio ricordare che dall'entrata in vigore dalla legge del 2006 la polizia postale ha conseguito risultati importanti, riassumibili in 166 persone arrestate, circa 250.000 siti monitorati, di cui 154 attestati in Italia. Dall'emanazione del decreto, ossia dai primi di gennaio in avanti sono stati effettuati 8.264 monitoraggi, individuando 151 siti pedofili, segnalati alle competenti forze di polizia di altri Paesi; sono state tratte in arresto 19 persone e denunciate altre 192; sono state effettuate oltre 150 perquisizioni. Naturalmente, questa normativa va integrata con uno sforzo che bisogna fare a livello europeo. Si tratta cioè di creare, come si dice in gergo, una sorta di *black list*, di lista nera europea di siti, in cui si possa intervenire a livello europeo con una cooperazione tra le diverse polizie. Io stesso ho incontrato, qualche settimana fa, il vice presidente della Commissione europea, onorevole Frattini, con il quale condivido la proposta, che lo stesso porterà avanti in sede di Commissione, per la creazione della suddetta suddetta *black list*, anche fornendo strumenti essenziali quali la tracciabilità dei pagamenti effettuati *on line* per l'acquisto di materiale pedopornografico ovvero - e su questo ho interpellato il collega Mastella - l'accesso ai casellari giudiziari per l'individuazione di coloro che hanno già subìto condanne o sono stati inquisiti per reati di pedofilia, anche questo a livello europeo. di un fronte - lo ripeto - in cui l'Italia sta facendo la sua parte. Abbiamo uno strumento, nella polizia postale e delle comunicazioni, veramente molto efficace, ma non c'è dubbio che questa battaglia, ogni volta che viene combattuta, trova nuove difficoltà e se non si raggiunge questo livello di coordinamento, almeno sul piano europeo, sarà comunque sempre difficile. Si è affermato che, al di là della lotta specifica alla pedopornografia, abbiamo almeno altre due grandi questioni da tenere presente: la prima è quella del continuo aggiornamento delle regole e dei codici; la seconda è quella dell'educazione, dell'informazione e del coinvolgimento delle scuole e delle famiglie. Dal punto di vista dei codici e delle regole, stiamo lavorando per per estendere alcune esperienze positive che abbiamo fatto in questi anni, penso ad esempio all'esperienza del Comitato "TV e minori" che, in un ambito situazione è certamente più agevole perché è molto più facile monitorare i programmi televisivi che non miliardi e miliardi di pagine Internet, ha ottenuto dei risultati.

con una particolare attenzione a un codice di protezione su Internet. Il lavoro è stato avviato innanzitutto con gli operatori, con gli Internet *service provider* e con gli operatori di telefonia, perché è chiaro che avremo sempre più la connessione a Internet a banda larga non non soltanto dai nostri PC, ma dai telefoni mobili. Se non ci saranno meccanismi di *parental control*, ossia di intervento per escludere per i minori la possibilità di accesso a Internet attraverso la telefonia mobile, che stiamo negoziando con le aziende di telecomunicazione, è evidente che l'accesso a Internet diventerà molto meno regolabile che non quello attraverso il *computer* di casa propria per una famiglia. Il lavoro di questo codice, che quando verrà definito passerà ovviamente in Parlamento per il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia, di cui alla legge n. 451 del 1997, è abbastanza avanzato. Direi che il codice si baserà sul concetto di tenere assieme la funzione importantissima di Internet per lo sviluppo mentale, informativo, culturale dell'infanzia e, al tempo stesso, la possibilità di forme forme di intervento e di controllo, sulle quali però - ed è l'ultimo tema su cui voglio soffermarmi - c'è bisogno certamente di un impegno della scuola e della famiglia più forte di quello che si è realizzato finora. Vedete, l'esempio è semplicissimo; come ho detto prima, abbiamo in casa, e avremo sempre più anche su un terminale mobile, la possibilità di accesso a miliardi e miliardi di pagine di informazione: grande opportunità, grandissimi rischi. Per gestire tale accesso è naturale che le famiglie e le scuole debbano condurre i bambini e i minori a conoscere, a frequentare e ad abituarsi all'uso della Rete. Non è facilissimo in questa prima fase, perché talvolta i genitori conoscono la Rete meno dei loro figli. Sarebbe come, per fare un esempio della mia generazione, se i miei genitori mi avessero

Credo che occorra, da questo punto di vista, un impegno straordinario delle istituzioni. Non è un impegno che grava solo sul Ministero delle comunicazioni, ma dev'essere assunto a livello intergovernativo. L'ultima legge sulla censura cinematografica, che contiene un capitolo sui videogiochi, prevede, ad esempio,

Lo dico nella consapevolezza di quanto sia delicato parlarne in giornate che procedono la finanziaria, ma del resto è anche il momento giusto per farlo. Nell'ambito delle proposte che il mio Ministero ha avanzato per la finanziaria, c'è anche quella di istituire

alla legge medesima, che hanno arricchito e ulteriormente rafforzato la tutela dei minori. Gli stessi provvedimenti del Governo vanno in questa direzione. È importante che il Paese sia unito nel tutelare l'infanzia e l'adolescenza dalla pedopornografia. È un aspetto importante che rende forte il nostro Paese; la nostra legislazione è stata ritenuta dal Comitato minori dell'ONU all'avanguardia nel mondo. Proprio nelle ultime settimane, il Governo italiano ha agito perché a Lanzarote, nella risoluzione del Consiglio d'Europa, venisse inserito il tema della protezione dei minori dalla pedopornografia. Sarebbe importante a tal proposito, proprio sulla base del lavoro che il Governo sta svolgendo e che va rafforzato anche con finanziamenti adeguati, che il nostro Paese accogliesse un convegno mondiale,

oggetto di grandissima attenzione da parte dei *media*, ma non sono poi soggetto di attenzione nella loro vita. Ci sono tante storie sui bambini, ma poca conoscenza sulla vita dell'infanzia e dell'adolescenza. Ma questo è un compito di tutti e la Commissione bicamerale per l'infanzia sta conducendo una indagine conoscitiva a cui inviteremo il Governo, che ha già dichiarato la sua disponibilità.

di tecniche e interventi per le scuole e le famiglie. Sarebbe stato molto opportuno se questa iniziativa fosse stata presa e gestita dal suo Ministero, magari insieme con il Ministero della pubblica istruzione perché poteva costituire una fonte di ulteriori conoscenze ed anche un *input* per ulteriori studi sia nelle scuole che nelle famiglie stesse che volessero approfondire l'argomento. Ma, a prescindere da questo, anche il fatto che il Comitato "Internet e minori" sia stato soppresso a favore di un allargamento del Comitato "TV e minori" non mi sembra molto opportuno. Quest'ultimo Comitato, infatti, ha già molto da fare,

aspetto, a mio avviso estremamente importante (e credo sia stato saggio da parte sua prevederlo in questo modo), e cioè il coinvolgimento dei *provider* nella gestione di tutte le problematiche che la Rete

solo i siti registrati sui *server* italiani, ma dobbiamo collaborare a livello transnazionale per provare a prevenire, ancora prima che a reprimere. Io credo sia importante l'equilibrio che lei ha stabilito, perché dobbiamo

*privacy* e l'uso consapevole della Rete. Non ci sono scorciatoie, è giusto -, come ha affermato il Ministro - che si

Ringrazio il Governo per la risposta esaustiva che ha fornito. Valutiamo positivamente il decreto emanato dal ministro Gentiloni nel gennaio scorso e realizzato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per rafforzare la lotta contro i contenuti pedopornografici pedopornografici presenti in Rete e lo sfruttamento di minori attraverso Internet. Allo stesso modo, prendiamo atto positivamente dell'impegno ribadito in materia dai Ministri della giustizia dei Paesi dell'Unione Europea nella riunione svoltasi lo scorso maggio a Monaco di Baviera e tuttavia riteniamo che sia un preciso obbligo morale del Governo e del Parlamento quello di non abbassare la pressione nel perseguimento di questo orribile e ripugnante delitto. È proprio per tale motivo che intendo presentare al più presto un disegno di legge contenente disposizioni in tema di violenza sui minori, per intensificare l'intervento dello Stato in materia. Il provvedimento, tra l'altro, prevederà l'inasprimento delle pene stabilite dal codice penale per i reati relativi ad abusi sessuali in danno ai minori, l'inserimento di nuove fattispecie, come la sottoposizione ai minori di materiale pornografico, e la previsione di nuove norme, come quella relativa alla inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa.

Dopo 16 anni dalla sua morte, la Confindustria siciliana ha deciso di espellere gli associati che pagano il pizzo e non denunciano. La presa di posizione della Confindustria, che segue quella delle grandi organizzazioni del commercio, ha un significato importante e crea uno iato con quella organizzazione, che al proprio interno aveva imprenditori collusi, condannati per favoreggiamento e per concorso esterno in associazione mafiosa. Per evitare che si ritorni al passato, si richiedono condizioni di maggiore sicurezza per denunciare le richieste estorsive. Penso anche a nuove misure, quali: incentivare la denuncia; modificare la legge sugli appalti, escludendo dagli stessi le imprese coinvolte in fatti estorsivi; collegare le politiche di incentivazione creditizia, fiscale e previdenziale finalizzate all'opposizione al racket; rimpinguare i fondi antiusura; garantire mezzi e straordinari alle forze dell'ordine. In conclusione, ritengo che tutto ciò possa, unitamente ad una politica non collusa alla mafia, evitare l'affermazione e l'arricchimento di quelle imprese che vivono sul rapporto con la borghesia mafiosa, che dà vita a forme imprenditoriali parassitarie.

Recentemente, il nuovo direttivo di Confindustria regionale ha impresso una svolta netta alla posizione assunta in precedenza facendosi promotore e portatore intransigente della cultura della legalità e del ripudio assoluto di ogni rapporto con la mafia, anche di soggezione alla richiesta di pizzo. Si registra, altresì, la comparsa di imprese a capitale di origine mafiosa o colluse o contigue all'associazione criminale. Al di là delle solidarietà espresse,

Signor Ministro, per decenni, nonostante la riconquistata libertà, l'imprenditoria siciliana ma anche quella nazionale, salvo qualche rara ed eroica eccezione, ha sempre ben convissuto con il potere mafioso, all'interno di un rapporto che in zoologia si chiamerebbe di simbiosi mutualistica e che in giurisprudenza si chiama concorso di reato. Oggi le cose stanno cambiando. Dopo Libero Grassi e dopo il qualitativamente grande movimento dell'associazionismo antiracket costruito sulla geniale intuizione di Tano Grasso, non c'è più alcun alibi per nessuno, nemmeno per le associazioni imprenditoriali di categoria che si stanno svegliando - per essere benevoli - dopo anni di disattenzione e nemmeno per lo Stato, che deve impegnare risorse sempre più grandi per proteggere visibilmente, immediatamente ed efficacemente gli imprenditori che si oppongono al ricatto mafioso.

Signor Presidente, anch'io, come i colleghi che mi hanno preceduto, ritengo che in Sicilia stia succedendo qualcosa di importante e di significativo. L'Assoindustria siciliana ha deciso di espellere dall'organizzazione gli imprenditori che accettano di pagare il pizzo e che non denunciano gli estortori. Singoli imprenditori si sono rifiutati di soggiacere al racket delle estorsioni e, seppure oggetto di attentati ai loro danni, hanno denunciato ed identificato gli estortori stessi. Essendo noto il rapporto stretto tra legalità e sviluppo, chiedo di conoscere la posizione del Governo e quali orientamenti e impegni il Governo intende assumere, già a partire dall'incontro che dovrebbe svolgersi il 3 ottobre prossimo venturo, per sostenere questa nuova nuova fase così importante e con quali strumenti ed iniziative il Governo intende dare attuazione alle proposte contenute nella risoluzione di maggioranza in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per quanto riguarda la Sicilia ed il Mezzogiorno.

il ripudio verso le organizzazioni mafiose ed un impegno collettivo, per l'appunto corale, perché i legami con il sistema imprenditoriale siano spezzati e venga meno la capacità della mafia, che purtroppo

un'articolata riflessione svolta dal Ministero dell'interno, voglio evidenziare che la strategia di Cosa Nostra consiste ancora nella ricerca della mediazione, nella capacità di inserirsi in modo efficace e silenzioso nei meccanismi economici, sia laddove ciò avviene

Una delle principali caratteristiche di evoluzione del fenomeno è legata alla presenza di soggetti dotati di un profilo culturale adeguato - operatori economici e finanziari - per sostenere una direzione dinamica di infiltrazione nell'economia.

l'avvicinamento di imprenditori formalmente estranei al sodalizio mafioso innesca, laddove si realizza, un meccanismo di reciprocità che garantisce a quegli imprenditori vantaggi non altrimenti conseguibili e alla mafia l'opportunità di allargare il proprio condizionamento verso settori dell'economia. Si deve, dunque, agire dal lato della repressione e da quello della prevenzione dell'infiltrazione. Anch'io sottolineo il particolare valore,

l'obbligo di denunciare i tentativi di estorsione, collusione e ricatto da parte delle cosche e di prestare collaborazione alle forze dell'ordine. Credo sia un fatto naturalmente importante, che si aggiunge anche ad altri codici etici via via assunti dalle organizzazioni di imprese.

meccanismi che governano, attraverso la stazione unica appaltante, un processo di unificazione e concentrazione degli appalti per fornire un contributo alla deterrenza

di meccanismi di collaborazione nuovi. In particolare, nell'accordo siciliano c'è il coinvolgimento delle banche, di Banca d'Italia e così via, per cercare di dare sostegno ed assistenza agli imprenditori che hanno avuto ed hanno problemi di racket.

L'obiettivo prioritario del piano, in questi anni, è stato quello di garantire un'integrazione con le componenti della sicurezza; si sono utilizzate figure di prefetti coordinatori, si è cercato di allestire un meccanismo di verifica anticrimine degli investimenti, di modo che l'informazione corresse verso gli enti locali, le istituzioni, le stazioni appaltanti e da parte degli organismi preposti alla sicurezza nel caso di segnalazioni utili a prevenire la presenza di soggetti mafiosi. Le Regioni hanno variamente allestito accordi di programma sulla sicurezza; cooptazioni, attraverso protocolli di legalità, degli attori della sicurezza; protocolli d'intesa con la Guardia di finanza; la Regione Sicilia ha predisposto un programma di questo genere. Dal punto di vista finanziario, della spesa e dell'allestimento di questi interventi, possiamo dire che il risultato è positivo, che i soldi sono stati spesi.

lo sviluppo avviene attraverso il diritto di cittadinanza, dove sta bene un cittadino in chiave di libertà, dignità e sicurezza, sta bene anche un'impresa in chiave di dignità, libertà e sicurezza. Pertanto, daremo la priorità al potenziamento dei servizi di base e delle condizioni di vita civile nel Mezzogiorno e al suo interno daremo molto rilievo al tema della sicurezza. Non elenco i sottotitoli di questo programma perché sarebbe troppo lungo, ma voglio dirvi solo che in sostanza l'oggetto è la sicurezza nel presidio del territorio e la diffusione della legalità per quel che riguarda, ad esempio, azioni di tutela del lavoro regolare, il contrasto del racket, la trasparenza degli appalti pubblici, con interventi che riguardano le tecnologie,

bisogna che portiamo la nostra discussione non sempre sul quanto, perché i soldi ci saranno e non sarà un miliardo in più o in meno, quando si parla di 100 miliardi di euro in sette anni, a cambiare il corso delle cose; a cambiare il corso delle cose sarà il come, come stavolta realizziamo questa operazione. Allora, comincio dicendo che già da questa finanziaria tutti i sistemi di incentivazione andranno via al massimo dall'intermediazione amministrativa e si metteranno in condizione massima di automatismo e di garanzia per chi deve approcciarli.

Lei parlava di sicurezza nel territorio, di libertà e di dignità; il racket è controllo del territorio - di questo c'è consapevolezza in questo Governo, anche per quello che stanno facendo i Sottosegretari competenti - ed è fonte di liquidità per la mafia, ma è anche gestione diretta delle imprese che da pulite diventano, in poco tempo, a gestione mafiosa. Ciò è dovuto anche ai tempi della giustizia, che devono essere sicuramente accelerati. È certo,

denuncia e alla partecipazione a gare di appalto per coloro che sono affrancati da questo tipo di meccanismo possano essere essenziali. Non è facile denunciare il racket, mettersi contro un mafioso o una cosca nel territorio del Sud, nella nostra terra

all'allontanamento di una clientela assidua da quello che può diventare un potenziale bersaglio della criminalità organizzata. Rispetto a tutto questo c'è bisogno di un maggiore impegno anche da parte delle forze dell'ordine che necessitano certamente di finanziamenti significativi anche in termini di mezzi e soprattutto di

Signor Ministro, prendo atto delle sue parole, ma temo che ci troviamo ancora sul generico e ci si riferisca a protocolli, a patti, a stazioni appaltanti già realizzati nella scorsa legislatura.

non ci entrava; oggi lì c'è la camorra in assenza del lavoro. Il problema allora si pone non solo e non tanto sotto il profilo della sicurezza perchè quando intervengono i magistrati e le forze dell'ordine il danno è già stato fatto, c'è già la mafia. Si tratta allora di convogliare al Sud investimenti, denaro che crei le infrastrutture e che incentivi l'impianto delle imprese, ovviamente con quei controlli qualitativi per evitare che poi si impiantino anche le imprese colluse e che il denaro finisca nelle

vede uno spostamento di investimenti verso il Centro-Nord e faccio presente che, nella scorsa legislatura, con la presenza nella compagine governativa di un partito a forte caratterizzazione settentrionale, ciò alla fine non si era verificato nella misura così rilevante con cui si sta manifestando oggi. un problema ulteriore, quello della diminuzione di fondi per il Ministero dell'interno. Noi non vogliamo l'Esercito; vogliamo più uomini delle forze dell'ordine che però intervengono in una situazione che è ormai diventata problematica. Infine, non vogliamo più eroi tra gli imprenditori, i sindacalisti, i cittadini. Dobbiamo fare in modo che non abbiano la pistola puntata alla tempia perchè, mi creda, signor Ministro, sarà difficile scegliere tra una pistola puntata alla tempia e l'essere buttati fuori dalla categoria produttiva di appartenenza. lavoro, lavoro, lavoro; creare investimenti e far sì che la cultura della legalità impartita nelle scuole possa trovare fuori la giusta applicazione. [DI

che mi convince abbastanza. Voglio preliminarmente spezzare una lancia a favore dell'imprenditoria siciliana. In realtà, poi, storicamente - basta vedere i processi tutti i grandi lavori, tutte le grandi progettazioni sono stati pensati negli studi di Milano. Le grandi società, da quelle del Vaticano, a quelle emiliane o piemontesi

la visione plastica dell'imprenditore al quale è stata bruciata l'azienda o che è stato minacciato che però, il giorno dopo, si riaffaccia sul suo territorio e ricomincia a lavorare rappresenta un'importante opera di propaganda contro la mafia e anche una grande opera di dissuasione.

Concordo con lei quando afferma che non è possibile garantire condizioni di adeguato sviluppo economico nelle aree in cui non si garantisce legalità e sicurezza e che quindi gli investimenti in legalità e sicurezza sono la precondizione per creare e sostenere lo sviluppo.

che nel Documento di programmazione economico-finanziaria che il Senato ha approvato con la risoluzione di maggioranza vi è una indicazione precisa, tendente a trasformare gli incentivi, ad esempio della in credito automatico di imposta per investimenti e occupazione. Mi pare questa un'indicazione importante, che sarebbe necessario che il Governo confermasse come orientamento, anche perché sono un po' preoccupato, di contro, nel sentire che si ipotizzerebbe la trasformazione di tutto il sistema degli incentivi semplicemente per riduzione degli utili di impresa, il che costituirebbe per il Mezzogiorno e per la Sicilia un ulteriore problema, certamente non un vantaggio. Per quanto riguarda la necessità che la Sicilia e il Mezzogiorno siano sostenuti nel loro sviluppo, utilizzo le affermazioni del governatore della Banca d'Italia Draghi, il quale sosteneva che non è possibile consentire al Paese Italia di crescere, se non cresce, appunto, il Mezzogiorno e quest'ultimo non può crescere, come abbiamo detto, se non si creano le condizioni di legalità e di sicurezza che ne consentano la crescita. Spero tutto quel che lei ha detto sia tutto, presto e bene, realizzato a partire dai prossimi provvedimenti che saranno al nostro esame, prima tra tutte la legge finanziaria e i provvedimenti collegati. Ringrazio i colleghi per le importanti sollecitazioni effettuate e per gli impegni assunti dal Ministro nel contrasto alla mafia in Sicilia e a difesa della imprenditoria siciliana.

signor Ministro, l'11 settembre scorso l'amministratore delegato dell'ENEL Fulvio Conti ha lanciato un allarme, subito raccolto dai *media**,* dicendo che siamo ancora a rischio di rimanere al freddo e al buio a causa di un elevato consumo di gas cui non corrisponderebbero scorte sufficienti. Vorremmo sapere se il Governo ritiene che esista un rischio sicurezza per il sistema energetico italiano e quali sono le misure e gli orientamenti che intende adottare in materia di energia.

come è stato accennato dalla collega senatrice appena intervenuta. Le chiedo quali iniziative a breve, signor Ministro, intende porre in essere onde escludere questo rischio che - sottolineo - è stato accentuato dal fatto che il suo Governo, in particolare il Ministro dell'ambiente, impedito l'utilizzazione di sovrappressione ai campi di stoccaggio in due località (una è a Settala, l'altra è a Fiume Treste) che invece

aumenti delle tariffe di gas ed elettricità; aumenti che non sono giustificati dall'aumento del prezzo del petrolio giacché le multinazionali del prezzo del petrolio sono dotate di scorte accumulate con dei prezzi solo per loro più favorevoli e quindi questo automatismo è ingiustificato ed inoltre hanno profitti in crescita. Altro elemento per la mia domanda è questo: finalmente in finanziaria vedremo porre fine alla scandalosa vicenda dei CIP6, che ha distolto risorse dalle fonti rinnovabili ed è tanto costata agli utenti. Il Governo deve investire sull'efficienza energetica, sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e per questa via intervenire sui costi dell'energia ai consumatori. Quali misure strutturali - e non parlo degli incentivi per i frigoriferi vecchi - vorrete assumere per coniugare insieme salvaguardia dell'ambiente, riduzione dell'emissione di anidride carbonica e sviluppo economico buono del Paese?

nell'attuale scenario di riduzione degli stoccaggi di gas, di congelamento dei progetti per gli impianti di rigassificazione, di rifiuto delle centrali a carbone pulito e del generale immobilismo dimostrato dal Governo nel trovare soluzioni concrete contro l'assoluta dipendenza del Paese dal gas o dall'energia elettrica francese, qual è la politica energetica del Governo che fino ad oggi non è stata peraltro messa in atto in risposta al contemporaneo aumento dei consumi energetici del Paese, al costante aumento del prezzo del petrolio ed all'allarme dei cittadini, soprattutto quelli del Nord, per i pericoli di *blackout* invernali, anche in considerazione del rinnovato interesse della Comunità Europea per il finanziamento di ricerche a tecnologia avanzata nel settore dell'energia nucleare, di cui altri Paesi intendono incrementare la produzione,

Signor Ministro, anch'io, con poca fantasia, mi rifaccio alle dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'ENEL, ma credo che abbiano particolarmente colpito. Tralascio quanto hanno detto i colleghi e riprendo soltanto quanto affermato oggi dall'amministratore dell'ENEL in un'intervista ad un quotidiano, richiesto al Governo un piano energetico incentrato su carbone e nucleare. Avendo pur presente il quadro di estrema debolezza in cui versa il nostro Paese, in una condizione di dipendenza storica

di ascoltare parole chiare e io mi propongo di dirle: il maggior elemento di criticità del fabbisogno energetico a breve l'approvvigionamento di gas naturale. Questo è il nostro problema al momento. Il nostro sistema di gas naturale è in condizioni di potenziale criticità (lo dico più popolarmente: "viaggiamo al pelo") dal 2004.

Credo, per quanto dirò adesso, che potremo uscire da questa criticità alla fine del 2008, se non intervengono fatti che oggi non riusciamo a valutare.

derivano dal fatto che stiamo andando a gas per produrre energia elettrica ormai per il 60 per cento della nostra produzione. È una tendenza che interessa tutti i Paesi d'Europa, ma noi siamo molto più su.

tutto qui. Adesso, per rimettere in moto queste operazioni molto complesse ci vogliono due o tre anni. Dall'altro Dall'altro lato, i nostri giacimenti nazionali sono in via di esaurimento e quelli nuovi non riusciamo a metterli in produzione per ragioni ambientali, autorizzative, di volontà locali e via dicendo.

la produzione idroelettrica ha avuto scarsi apporti naturali con i bacini ghiacciati e poi poca neve quando era il momento. Quindi, scarsa produzione.

devo dire sinceramente che mi riserverò via via di estrapolare qualche misura; lo dico molto sinceramente per senso responsabilità, per il dovere che mi compete e per la preoccupazione che certamente ho sulle prospettive della sicurezza del sistema. Abbiamo promosso, avviato e spinto il potenziamento dei tubi, pensiamo ai tubi che arrivano dall'Austria (qui c'è qualche problema, ma una prima parte di potenziamento si concluderà) e a quelli che arrivano dalla Tunisia e

Il punto cui lei, senatore, faceva riferimento riguarda il potenziamento di uno stoccaggio che è stato inibito da questioni ambientali. Io sto discutendo con il collega Pecoraro Scanio per trovare una soluzione,

non vorrei che si diffondesse anche sugli stoccaggi una psicologia negativa. Laddove ci sono dei buchi, che ormai sono vuoti, fa bene metterci dentro qualcosa

Abbiamo fatto accordi con Austria e Albania per dei cavi elettrici; stiamo lavorando con il Montenegro. Insomma, stiamo cercando di sviluppare una strategia, recuperando iniziative già avviate con il precedente Governo, portandole avanti, aggiungendone di nuove.

alcune misure, quali l'obbligo di massimizzare le importazioni di gas, misure per il risparmio incentivato con premi e penali per le imprese che consumano gas, faremo una campagna di informazione ai cittadini; siamo sempre in monitoraggio.

riguarda il tema dell'energia in Italia, che costa tantissimo rispetto ad altri Paesi. Il costo è alto per vari motivi, compresi quelli del *mix*.

Questo è evidente, ma il meccanismo di regolazione dei prezzi non può non fare riferimento al petrolio, tanto è vero che la nostra Autorità per l'energia si comporta in questo senso. Naturalmente il *mix* che abbiamo noi costa molto caro, questo va da sé. Come vogliamo e possiamo riequilibrarlo?

attuali non ritengo credibile - so che è oggetto di discussione - lanciare un piano nucleare a questo livello di tecnologia in Italia, non solo perché facciamo fatica anche a localizzare un sito provvisorio di deposito, ma anche

dobbiamo inserirci credibilmente nella ricerca nucleare di quarta generazione, quella cioè che sostanzialmente si propone di risolvere il problema delle scorie, che ha alti meccanismi di sicurezza intrinseca, attrezzature ed altro. Credo che l'Italia debba rientrare in questo discorso di ricerca

le politiche di efficienza energetica, di risparmio energetico e di qualità ambientale possano effettivamente essere un volano della crescita ed avere una centralità nella crescita. Ciò significa però che tutte le culture ambientali e tutti coloro che hanno a cuore i problemi ambientali si rendano conto che vi è una razionalità del sistema che deve essere garantito. Se vogliamo andare a gas, che è il modo più pulito di produrre energia, dobbiamo avere almeno le infrastrutture per il gas. gas. Non sono accettabili posizioni che neghino questa verità, da qualsiasi parte vengano. Abbiamo bisogno di 2-3 gassificatori, dobbiamo potenziare 2-3 tubi e dobbiamo avere un po' di riserve dentro ai buchi

Penso che il tema dell'energia va a intersecarsi con questioni fondamentali anche di tipo economico, perché parliamo della competitività del nostro sistema economico. Come lei ricordava, le imprese italiane sostengono costi più elevati che nel resto d'Europa per l'approvvigionamento energetico. Si parla anche di sicurezza negli approvvigionamenti e di sostenibilità ambientale. Mi sento di condividere la scelta del Governo riguardo alla diversificazione delle fonti, con un *mix* energetico composto di gas, di carbone e di fonti rinnovabili, o anche scelte che ha prodotto proprio il suo Ministero sulla liberalizzazione del mercato, consentendo una competitività maggiore che dovrebbe portare all'abbassamento dei costi per i consumatori. A ciò si aggiunge anche una politica di misure per la sicurezza energetica, limitando i consumi e potenziando anche nuovi stoccaggi. incentivare, lo ha dichiarato prima riguardo all'esempio tedesco, le fonti rinnovabili, il fotovoltaico, l'eolico, le biomasse, anche se in questo scontiamo profondi ritardi. Concludendo, signor Ministro, anch'io, come lei, penso che non possiamo assolutamente uscire dal campo della ricerca internazionale, perché con essa garantiamo anche il futuro del nostro Paese

per garantire la propria sicurezza energetica. Lei faceva riferimento all'installazione di nuovi gassificatori che necessitano anche di una maggiore negoziazione sul territorio.

Segnalo che nel piano di assegnazione delle quote di immissione di CO2 nell'atmosfera c'è una penalizzazione esplicita degli impianti a carbone

È ora di fare il piano energetico nazionale per capire quanti buchi eventualmente bisogna riempire o se c'è proprio bisogno di gassificare. Vorrei

alla mercé di un'opinione, di una dichiarazione dei *media* e di un livello di informazione che trovo insufficiente. Il nostro sistema energetico è basato su combustibili fossili e ci costa caro, ma costa caro anche il nucleare. Leggevo che negli ultimi 30 mesi il prezzo dell'ossido di uranio che è fondamentale è aumentato del 670 per cento. Costa caro anche il carbone, carissimo visto quanto ne usano - ahimè - in India e in Cina.

Taglio. Ho parlato di aumenti dei costi per gli utenti. Non posso non ricordare il pensionato che è stato beccato qualche giorno fa a rubare per mangiare. Siccome

Vede, signor Ministro, nelle Aule parlamentari stiamo assistendo ad una totale ed arrogante chiusura al dialogo e al dibattito sulle fonti energetiche alternative a quelle tradizionali (vale a dire petrolio e gas),

soggette a continue oscillazioni di mercato, a continui aumenti. Notiamo che il Paese è carente (l'ha detto lei stesso) negli stoccaggi di energia, che c'è il pericolo di nuovi *blackout* e di fronte a questa panoramica abbiamo una parte del suo Governo (lo sa benissimo, purtroppo), le cosiddette correnti parambientaliste del suo

delle nuove tecnologie cui lei ha fatto riferimento. Si rifiutano di tener presente che il Paese, la nostra industria, oltre ad avere

di riuscire a portare a termine parte di quanto ha detto, ma le ripeto che con questa maggioranza, vista la protervia con la quale si preclude ogni discussione nelle Commissioni e nelle Aule, ho i miei dubbi che

ha detto. Soddisfazione e condivisione rispetto al messaggio più generale che manda al Paese. Credo che non siano utili le forzature che ha esercitato l'amministratore delegato dell'ENEL Fulvio Conti,

*(Ulivo)*. Signor Ministro, la recente impennata dei prezzi, non generalizzata, ma riferita in particolar modo ad alcuni generi alimentari di prima necessità, quali il pane, il riso, la pasta, i prodotti lattiero-caseari, la carne e la frutta, preoccupa e mette in difficoltà diversi consumatori e le famiglie, che non hanno visto crescere altrettanto celermente il loro potere d'acquisto. Inoltre, a seguito della forte riduzione dei consumi, compromesse la solidità di alcuni comparti della filiera agroalimentare e la stessa redditività degli imprenditori del settore agroalimentare. Tenuto conto che il Governo ha già avviato iniziative concrete per approfondire e portare a soluzione tali problematiche (penso al tavolo di confronto tra consumatori e commercianti, l'osservatorio prezzi e tariffe del Ministero dello sviluppo economico), chiedo di sapere se il Governo intende adottare ulteriori iniziative per contrastare gli aumenti ingiustificati e in alcuni casi speculativi dei prodotti alimentari.

in particolare climatici, sia a fattori strutturali. Uno dei fattori strutturali, che ha provocato un notevole

è una misura drammatica per la nostra economia, che non potrà che avere gravi riflessi in termini di aumento dei prezzi delle derrate alimentari. Vorrei sapere se lei condivide questa misura.

ma parliamo del piatto di pasta, quello più semplice con il sugo di pomodoro, del mezzo bicchiere di vino, della fettina di carne e della mezza pagnotta, cioè di quei prodotti che, in compagnia di poco altro, riempivano, fino a poco tempo fa, la sporta della signora che andava a fare la spesa; oggi riempiono lo *shopper*, un termine inglese che sta ad indicare quella indicare quella busta di plastica che i pensionati e le pensionate utilizzano per portare via la spesa quotidiana.

a ragioni strutturali, a politiche agricole ed energetiche, a modelli di distribuzione, a modificazioni climatiche. Quali strumenti sono stati adottati per fronteggiare l'emergenza? Qual è il livello di attenzione al riguardo? Quali ricadute su questa dinamica dei prezzi hanno quei grandi processi ai quali facevo riferimento, molti dei quali ricadono anche

possa registrare dal lato dell'andamento dell'inflazione qualche segnale di crescita proprio per questo tipo di prodotti. Certo l'origine del problema è da attribuirsi a questioni strutturali, a quotazioni dei prezzi delle materie prime

stiamo proponendo all'Unione Europea, come stanno facendo anche altri Paesi, l'immediata estensione delle superfici coltivate a frumento per il prossimo anno e l'avvio di una discussione anche per quanto riguarda il latte, al fine di ottenere una produzione più ampia e quindi evitare tensioni sui prezzi. Abbiamoconvocato i rappresentanti del commercio per discutere i fattori di criticità di alcuni mercati, che abbiamo anche

Inoltre, c'è un rafforzamento dei meccanismi di osservazione. Abbiamo rafforzato l'Osservatorio prezzi e rilanciato il sito apposito. Oggi un cittadino può verificare direttamente il livello minimo, medio e massimo dei prezzi al consumo di un paniere di 66 beni di largo consumo in 38 capoluoghi di Provincia. Aggiungo che stiamo realizzando con InfoMercato un'operazione su 15 piazze italiane, che sta registrando tutti i prezzi di alcuni prodotti di base, a cominciare dagli ortofrutticoli, dei mercati all'ingrosso e saremo in condizioni di rilevare in tali mercati anche i rispettivi andamenti dei prezzi e le diverse situazioni al dettaglio. Vedremo poi nei limiti, lo chiederemo all'*antitrust*, che uso fare di questi dati; tuttavia, il sistema di informazione si sta notevolmente potenziando.

le anomalie di prezzo che riscontrassero sui territori; abbiamo quindi messo in rete i dati delle Camere di commercio e ho firmato - adesso è alla controfirma del ministro Padoa-Schioppa - una nuova convenzione con la Guardia di finanza

allora c'è poco da fare. Ci vuole consapevolezza che su tali questioni non si scherza e che a nessuno è consentito - a chi pratica commercio, intermediazione, eccetera - ritenere che un centesimo non valga nulla, perché nel sistema questo meccanismo ci porta fuori limite. Infine, siccome so che al pensionato che si trova il pane a tre euro, non gli puoi dire che hai risolto con la ricarica del telefonino, affermo anche che dobbiamo operare il massimo sforzo - abbiamo cominciato a farlo adesso con il protocollo firmato e ad ottobre ci sarà nelle tasche di alcuni pensionati qualche primo risultato, ma dovremo continuare anche in questa finanziaria rimboccare i livelli di reddito delle condizioni più basse. Questo è un punto che io credo venga prima

ma anche la complessità di questo tema che sovrappone - come si diceva - elementi diversi: fattori congiunturali legati anche alla produzione delle materie prime, fattori strutturali, che già anche altri colleghi richiamavano e, quindi, una nuova dinamica dei mercati internazionali, una domanda che cresce, effetti anche delle riforme delle politiche europee che giustamente, a mio avviso, debbono anche rivedere, alla luce di questo nuovo scenario internazionale, le dimensioni produttive dei singoli Paesi e, quindi, anche delle nuove dinamiche. Credo che a maggior ragione il nostro Paese, proprio per questo movimento che c'è rispetto ai mercati internazionali, agli effetti anche delle importazioni e delle esportazioni, debba tenere conto degli elementi che lei diceva. Da una parte, un un enorme rigore per quanto riguarda l'osservazione e il controllo e, in qualche modo, l'autoregolamentazione del settore per quanto riguarda i prezzi, e dall'altra, ritengo che questa sia una risposta più strutturale e non immediata, ma assolutamente esigente, di una riorganizzazione del nostro sistema dell'offerta. Ricadiamo sempre nel problema della grande

anche le sue manifestazioni di rispetto nei confronti del mercato. L'espressione *moral suasion* è quella più indicata per evitare che si prendano a pretesto

di contribuire efficacemente alla prosecuzione ed al rilancio di quei risultati positivi che in questo primo scorcio di attività governativa sono stati conseguiti nel rilancio dell'economia. Credo che questa sia una condizione indispensabile e fondamentale alla quale non possiamo assolutamente sfuggire.

della questione del modello energetico e delle politiche europee. Credo che dobbiamo compiere lo sforzo di mettere in relazione le ricadute che si hanno su queste questioni che hanno così rilevanza sociale con le scelte operate a livello sovranazionale complessivo, perché così potremo mettere sulla bilancia anche questi elementi con le conseguenze dell'impazzimento del clima, con i costi della inazione su tutta una serie di terreni, con le scelte energetiche e con il governo complessivo dell'economia.

le competenze del Governo siano ristrette per intervenire su questa materia, ma credo che quelle che ha messo in campo siano azioni efficaci, che hanno prodotto anche risultati, tenendo conto che siamo in un sistema di mercato libero e aperto.

che lei abbia detto che anche nella prossima legge finanziaria ci sarà una particolare attenzione alla necessità di far recuperare reddito e capacità di potere d'acquisto alle fasce più basse, perché credo che alcune siano veramente in condizioni che posso definire drammatiche.